nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. Ha la parola il senatore Buccarella per illustrare la richiesta. siamo qui a illustrare la richiesta di procedimento d'urgenza prevista dall'articolo 77 del Regolamento che

nel 2015 è stata approvata la cosiddetta legge anticorruzione, che il mio Gruppo non ha votato perché, anche in seguito a una consultazione *on line*, avevano in essa notato molte pecche. Non era prevista l'estensione del cosiddetto DASPO per i corrotti, e cioè la previsione di interdizione perpetua dai pubblici uffici

l'Assemblea non si vorrà lasciar sfuggire. Si tratta della previsione di una figura investigativa, di un mezzo preventivo per battere la corruzione, che è l'utilizzo dell'agente sotto copertura o agente infiltrato per i reati contro la Iniziamo con il dire che si tratta di una figura non nuova che noi vorremmo istituire, ma che è già presente da dieci anni nel nostro ordinamento, con la legge n. 146 del 2006, e che noi vorremmo integrare prevedendo l'utilizzo di agenti di polizia giudiziaria indagini preliminari già avviate, sotto la direzione di una procura, da infiltrare per

non su elementi di fatto. Qui non si parla dell'agente provocatore. Noi non vogliamo inserire una figura che istiga al reato promettendo o dando mazzette a questo o a quel pubblico ufficiale. Cortesemente, quindi, eventuali interventi successivi facciano a meno di criticare la nostra proposta facendo riferimento a questa figura, che pure esiste in altri ordinamenti giuridici ma di cui qui adesso non si sta parlando. Stiamo parlando non dell'agente provocatore,

immettere immagini pedopornografiche, ma semplicemente inserendosi nel flusso, soprattutto telematico, di Internet agiscono e, fortunatamente, costantemente scoprono

fatti, difficilmente l'autorità giudiziaria, in esito a dei giudizi, può pervenire a sentenze di condanna o assoluzione perché la prescrizione

o per altre casualità che vedono emergere il fenomeno corruttivo a distanza di molto tempo. Ribadisco che gli agenti sotto copertura

molti magistrati e operatori di prima linea che, in varie occasioni, hanno espresso il loro favore per l'introduzione di questa figura, a partire dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, fino all'attuale presidente dell'Associazione nazionale magistrati, al procuratore di Roma e tanti altri. Noi non vogliamo farci necessariamente forti di pareri che, per quanto autorevoli, sono sempre pareri e quindi opinabili. Vogliamo invece impostare il discorso su criteri oggettivi, chiedendoci cioè se oggi il Senato non ritiene opportuno velocizzare l'*iter* legislativo per far sì che l'agente sotto copertura per i reati di corruzione sia finalmente introdotto in Italia. Noi siamo convinti che la maggior parte dei nostri cittadini, a prescindere da come votano, sia del nostro stesso parere e ci auguriamo anche del vostro. Speriamo,

a queste misure anticorruzione. È questa un'altra splendida occasione per dimostrare che la politica dei partiti non è quella rinunciataria e del no finalmente trovare insieme su qualcosa in comune che non possiamo non condividere. Per questo motivo chiedo il voto favorevole all'Assemblea e speriamo bene, insieme a tutti gli italiani, che questa misura sia adottata e il suo *iter* sia velocizzato.

l'argomento è molto fascinoso, ma farei una distinzione tra merito e provvedimento d'urgenza. Va da sé che ci troviamo in una situazione estremamente delicata, nella quale viviamo la difficoltà se il provvedimento d'urgenza, come io mi auguro

Credo, però, che la richiesta che il Movimento 5 Stelle avanza sulla necessità di creare una via prioritaria per iniziare a discutere dell'argomento possa essere francamente

Innanzitutto, come ho già detto l'altro giorno, bisogna che ci mettiamo d'accordo sulla diagnosi: secondo i dati forniti dalle associazioni che combattono siffatti fenomeni, sono circa 9 milioni gli italiani che ogni anno si sentono chiedere una tangente - andate a vedere sui siti le percentuali

e non di un esame del fenomeno, che è da combattere e reprimere dal punto di vista penale, senza però arrivare a soluzioni come quelle

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale - esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - non è comunque punibile - colleghi, un po' di attenzione, perché, quando capiterà a voi di incappare in norme di questo tipo, sarà tardi per chiedersi cosa stia succedendo

altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi». Chi conosce un po' la storia d'Italia - porto solo due esempi eclatanti, che interessarono anche nostri colleghi parlamentari, che prima erano stati magistrati - ricorderà i fatti di Genova:

di preparazione del reato o di partecipazione materiale alla sua commissione erano determinati dal fatto che egli stesso, sotto copertura, intendeva smantellare la banda di trafficanti di droga.

dopo processi, processi e processi di assoluzione c'è ancora chi insinua che il generale Mori, nelle sue indagini contro la mafia, abbia operato in una determinata maniera non per combattere la mafia, ma, viceversa, per fini

che, giustamente, magari fingendosi impiegati del catasto, ingegneri di opere pubbliche o in qualsiasi situazione in cui si muovano i pubblici dipendenti o i pubblici ufficiali, vengano a

con grande disprezzo per le garanzie delle persone, per raggiungere un obiettivo, calpestavano i principi fondamentali di uno Stato democratico. Un meccanismo di questo tipo, lungi dal risolvere i problemi della corruzione, introdurrebbe altre tossine nel corpo dell'ordinamento, creando un immenso polverone, all'interno del quale colpevoli, innocenti, persone indotte o che simulino di che simulino di accordarsi per commettere un reato, anche se non lo commettono, oppure che partecipino materialmente alla sua commissione, creano sicuramente, a livello di processo, un ginepraio:

«nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero (...)». Ci mancherebbe altro che non fosse nell'ambito di un'indagine e su delega del pubblico ministero, e cioè che l'agente provocatore sotto copertura pensasse da solo di svolgere questa attività senza che nessuno glielo chieda, cioè che ogni maresciallo dei carabinieri e ogni questura pensasse da se di infiltrare persone all'interno degli uffici pubblici dei Comuni con il compito di simulare o commettere reati per poi incastrare

il fatto che persone che fanno parte degli uffici possano denunciare un fatto mi sta bene e anche questo lo dirò in ogni trasmissione televisiva. Un conto è essere all'interno di una certa realtà e venire a conoscenza di situazioni di malaffare in corso o

ha generato poi, nella sua applicazione, una disomogeneità sul territorio, sia nelle azioni di prevenzione e di controllo che nei processi autorizzativi. Questo è accaduto per vari motivi noti, ma anche e soprattutto per le evidenti differenze negli stanziamenti dedicati sia in risorse finanziarie che in personale. La fotografia che oggi abbiamo ritrae un Paese che funziona con sistemi e velocità diverse e appare anche evidente la relazione tra i minori investimenti nel sistema della protezione ambientale e la presenza di gravi e dilanianti problemi per la salute dell'ambiente e delle persone. Sono emersi più esempi: ricordo tra tutti l'ILVA di Taranto e la terra dei fuochi. Quello che proponiamo oggi con il provvedimento in esame è un passo avanti verso una maggiore equità e una maggiore omogeneità nelle azioni di prevenzione e controllo, con l'obiettivo di livellarci all'asticella più alta sul punto della qualità dei comportamenti, delle prassi e dei risultati. È un obiettivo - lo sappiamo, bisogna essere concreti e reali - che ha difficoltà a convivere con quell'invarianza di spesa che abbiamo dovuto inserire. Come abbiamo detto, le differenze sono generate non solo, ma soprattutto da minori investimenti. Possiamo dire, però, di aver tutti insieme maturato questa consapevolezza e di essere pronti e impegnati per i passi successivi. Sempre legato al nodo dei finanziamenti è il tema della ricerca, che il sistema delle Agenzie-ISPRA svolge in modo complementare e coordinato. Naturalmente più riusciremo a garantire l'autonomia finanziaria del Sistema e più avremo garanzia di tutelare sia la ricerca, sia l'ISPRA dal rischio di un conflitto di interesse. *(Applausi dal Gruppo PD).*

ritengo che la proposta di legge all'esame dell'Assemblea vada a rafforzare il rendimento delle attività di protezione dell'ambiente, oggi devolute in modo frammentario a una pluralità di soggetti, in un'ottica di coordinamento sinergico fra questi ultimi e di un più efficace utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Questo disegno di legge si pone nel solco di una incisiva attività di modifica e innovazione in campo ambientale, avviata ormai da tempo dal Governo e dal Parlamento. È un tassello importante, che si aggiunge a un mosaico normativo che sta progressivamente prendendo forma dopo l'approvazione della legge n. 68 del 2015 (cosiddetta ecoreati) e l'introduzione di importanti novelle legislative previste dalla legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale). In tale contesto, il disegno di legge in esame persegue l'obiettivo di armonizzare e omogeneizzare le attività conoscitive e di controllo in materia di protezione ambientale, ad oggi attribuite a diversi soggetti. Tale volontà di rafforzare i momenti di coordinamento tecnico e di *governance* unitaria, tenendo comunque in considerazione gli ambiti di competenza dello Stato e delle autonomie territoriali, emerge con chiarezza dall'esame di specifiche disposizioni contenute nella proposta di legge. Due sono i punti che mi preme sottolineare. Vengono introdotti i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che dovranno fungere da parametri delle prestazioni delle Agenzie, e viene previsto un programma triennale delle attività del Sistema nazionale, che potrà conferire alle stesse maggiore organicità, favorendone la pianificazione in un'ottica di medio periodo. Permettetemi di porgere un sentito ringraziamento, oltre che ai senatori della Commissione ambiente, a ISPRA, nelle persone del suo presidente e direttore, alle singole ARPA e ai loro direttori, per il fattivo e costruttivo contributo che hanno dato a questo provvedimento. Non mi esimo dal rispondere anche alle critiche che sono state formulate in quest'Aula. Si poteva fare meglio, è stato detto, e questo sempre. Ma abbiamo scelto di portare a termine un provvedimento sul sistema delle Agenzie ambientali riteniamo sia fondamentale costituire lo strumento affinché sia garantita, su tutto il territorio nazionale, l'uniformità e l'adeguatezza degli *standard* di tutela ambientale.

GIARRUSSO *(M5S)*. Onorevoli colleghi, a nome del Movimento 5 Stelle chiediamo che il Governo venga a riferire in Assemblea, con la massima urgenza, sui fatti accaduti ieri notte in Sicilia. È soltanto per la grande professionalità delle Forze dell'ordine, colleghi, che oggi non siamo qui a commentare l'ennesima strage mafiosa.

Riteniamo che questo sia un fatto di una gravità assoluta, che testimonia il tentativo di rialzare la testa da parte della mafia tortoriciana, che in quei territori è ancora forte. Chiediamo che il Governo venga a riferire con la massima urgenza.

visto che il disegno di legge non lo riprende in modo strutturale, pur se presente nello stesso regolamento dell'ISPRA, che prevede l'attività di un Consiglio federale. Il disegno di legge al nostro esame cancella addirittura mentre noi riteniamo che il federalismo, anche nell'ambito dei controlli e dei monitoraggi ambientali, sia un punto di forza rispetto a un accentramento del sistema.

al Governo che, nelle funzioni di vigilanza svolte dal Ministero dell'ambiente, si preveda ad assicurare

apre una nuova finestra") *(M5S)*. Signora Presidente, intendo illustrare l'ordine del giorno G1.101, in quanto la maggior parte degli articoli contenuti in questo disegno di legge rinvia a successivi decreti attuativi. Di fatto si tratta di una disciplina non immediatamente esecutiva, ma che dovrà attendere l'adozione di successivi decreti di attuazione per essere effettivamente operativa.

venga fatto nei tempi più celeri possibile e preveda eventuali sanzioni per quei funzionari e soggetti della pubblica amministrazione che non adempiano nei tempi dovuti a effettuare l'emanazione di tali decreti attuativi.

a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in cui confluiscono: i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2, nonché dell'articolo 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

potrebbe essere anche la giusta specifica per i versamenti delle sanzioni amministrative che fanno riferimento, appunto, alle prescrizioni della parte sesta.

ordini del giorno a mia prima firma siano già stati accolti dal Governo, ma questo non ha comportato un'effettiva norma

tengo a ribadire che questo fondo, costola del Fondo unico giustizia, per tutte le parti che riguardano le sanzioni amministrative, i sequestri e le confische di sezioni ambientali non va incidere sull'equilibrio finanziario e quindi c'è invarianza finanziaria. A mio parere, quindi, potrebbe passare anche l'emendamento, dato che comunque, grazie all'emendamento del relatore in Commissione, dettato dalla Ragioneria di Stato, questo provvedimento dovrà comunque tornare alla Camera.

ci fu uno studio veramente eccezionale che stabilì cosa dovesse intendersi per «beni comuni». Mi ricordo anche che la campagna elettorale del denominata «beni comuni». In questo caso stiamo dando la possibilità al PD di far ricredere quantomeno quelle fasce della popolazione che possono aver inteso che ormai il ha distrutto la sinistra italiana. In questo caso, se volete rispettare quello che avete detto in campagna elettorale, ossia che volete realmente difendere i beni comuni, noi vi stiamo dando un *assist*. Potete, come risorgere. Quello che diciamo è che questo sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela

Quindi, chiedo al Partito Democratico di rispettare il patto con gli elettori, ossia quello che avete detto in campagna elettorale. Presidente, adesso lo vedremo dal voto.

Presidente, illustro l'emendamento 2.13 che vuole introdurre, all'articolo 2, tra le definizioni, l'«indice territoriale sintetico» quale parametro numerico calcolato in base alle caratteristiche significative dal punto di vista ambientale delle varie realtà territoriali e che vuole assegnare un peso ad ogni Regione in funzione della consistenza quali-quantitativa

quindi indispensabile inserire un principio di rappresentatività territoriale, peraltro, lo voglio sottolineare, riconosciuto anche a livello costituzionale. In sostanza, con questo indice territoriale sintetico abbiamo la presunzione di voler inserire un voto ponderale nel Consiglio - che noi continuiamo a chiamare «federale» - e proporzionale allo stesso indice territoriale sintetico.

in ordine alle richieste che ci vengono dalla Ragioneria dello Stato, è conforme. Io ribadisco, come ho già fatto prima (ma ci tengo a ripeterlo), che questa è l'occasione per dar seguito a quella che comunque è una volontà già espressa dal Governo: quella di costituire questo Fondo unico ambientale che da più parti è atteso e sollecitato.

al comma 2, specifica la finalità di questo Fondo: la prevenzione e il contrasto di condotte lesive dell'ambiente (e sappiamo quanto sia necessario e urgente), nonché la bonifica e il recupero dei siti inquinati. Quindi, ribadisco la necessità in questa sede di dare subito seguito alla volontà espressa dal Governo anche perché, con la votazione e l'inserimento dell'articolo 17 in Commissione, questo provvedimento - ahimè - tornerà comunque alla Camera, e se dovesse tornare con questo altro emendamento al suo interno, sarebbe cosa buona e giusta.

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire per assicurare un adeguato coordinamento tra il Sistema nazionale e le aziende sanitarie locali e le Forze di polizia di specialità al fine di realizzare la massima fruibilità delle informazioni in materia ambientale.

manca, a nostro parere, la valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio. Sappiamo che il sistema nazionale attualmente soffre di gravi squilibri territoriali quindi, ci si pone l'obiettivo di omogeneizzare e riequilibrare. Tuttavia, è anche importante che l'osservazione dei fatti porti alla valutazione delle necessarie azioni di riequilibrio e che, quindi, la funzione sia specificamente inserita nell'articolato

attribuisce al Sistema nazionale le attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse sia nazionale, che locale. Segnalo che l'azione di monitoraggio di una grande opera è normalmente posta a carico del suo realizzatore (si tratta di una prescrizione inserita nella pronuncia di compatibilità ambientale).

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede la collaborazione del Sistema nazionale con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché

opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di divulgare anche autonomamente programmi di educazione ambientale e di formazione in materia ambientale. un altro elemento di autonomia delle Agenzie rispetto a un'ipotesi eccessivamente centralistica. *(Applausi

alla lettera *c)* si parla di attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo; tale lettera conclude affermando che: «Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera

l'emendamento 3.211, il quale suggerisce che tra i compiti e le funzioni del Sistema nazionale sia inserita anche la definizione dei costi *standard* delle

indispensabile definire con attenzione costi che siano omogenei sull'intero territorio nazionale e che rispettino le realtà maggiormente virtuose. Infine, signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.26.

G3.107, proprio al fine di impedire la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree dove esiste già una notevole concentrazione di questo tipo di installazioni, quindi con un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante, si ritiene necessario e importante definire un indice di pressione ambientale. La normativa vigente, tra l'altro richiamata in questo ordine del giorno, attribuisce esplicitamente allo Stato la potestà esclusiva di individuare i criteri generali e le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione di questi impianti di smaltimento. Con l'ordine del giorno in parola chiediamo quindi al Governo di assumere ogni iniziativa necessaria, anche con atti normativi, a emanare un criterio che consenta di introdurre un limite di localizzazione delle discariche e delle fonti emissive in acqua, suolo ed aria legato in particolare alla saturazione del territorio, come l'indice di pressione ambientale. Per quanto giorno G3.108, si stima che nella Provincia di Brescia siano stati interrati complessivamente 35 milioni di metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non. Tra l'altro, il bresciano ospita i più importanti impianti per rifiuti pericolosi e la più grande discarica, che nel 2013 ha accumulato circa l'80 per cento dei rifiuti pericolosi dell'intera Regione Lombardia. Chiediamo quattro impegni specifici. Con il primo - che sicuramente troverà la contrarietà di questo Governo, che è a favore delle *lobby* dei petrolieri, degli inceneritori e dei grandi gestori di discariche - abbiamo chiesto una moratoria

punto - e spero che almeno su questo non vi sia il parere contrario - chiede che il Ministero si attivi con la Regione affinché quest'ultima possa dare tutte le informazioni necessarie ai cittadini, che sulla loro pelle

venissero messi a conoscenza di una situazione che è poco nota, quella del sito di interesse nazionale chiamato Caffaro. In quest'area, per decenni, vi è stato uno sversamento di PCB e di altri inquinanti da parte della azienda Caffaro, che è stato scoperto solo grazie ad alcune ricerche storiche e ad alcune analisi effettuate intorno al 2000. Sono passati circa sedici anni da allora ed è stato fatto poco o niente. Recentemente, il Ministro dell'ambiente ha dichiarato che

punto, di trovare i 42 milioni di euro promessi. Recentemente il nostro sindaco è andato dal Ministro e ha chiesto ulteriori risorse. Gli sono stati promessi - e solo promessi - ulteriori quattro milioni di euro: è un po' poco rispetto ai 42 milioni, che già sono pochi, per effettuare le bonifiche. Stiamo parlando di un'area di un'area in cui vi sono infiltrazioni nel suolo fino a 50-70 metri, un'area che è forse cento o mille volte (non è ancora ben definita la vera natura dell'inquinamento e la quantità

del Senato, impegna il Governo: ad intervenire affinché sia previsto il coinvolgimento del livello regionale anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» previsto all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge; a valutare l'opportunità di prevedere, alla luce degli inscindibili nessi esistenti tra ambiente, salute, sostenibilità e crescita, compatibilmente con l'equilibrio della finanza pubblica,

competenti; a garantire, anche valutando l'opportunità di ulteriori interventi normativi, che le attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica di ISPRA e delle agenzie siano svolte in maniera autonoma o in raccordo con altri soggetti istituzionalmente operanti nel settore della ricerca, a dotare il Sistema nazionale di ulteriori risorse al fine di implementare nel miglior modo possibile, su tutto il territorio nazionale, i servizi indicati, nonché a potenziare e coordinare le attività. nella materia ambientale, impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della presente legge, di assumere le opportune iniziative affinché sia assicurata la possibilità per le agenzie regionali di divulgare anche autonomamente programmi di educazione ambientale e di formazione in materia ambientale.

svolga anche attività di verifica sui monitoraggi che sono messi in campo dai soggetti privati che realizzano opere infrastrutturali, soprattutto a livello nazionale. mi sembra un impegno debole e quindi chiedo alla rappresentante del Governo, sottosegretario Degani, e alla relatrice di lasciare l'ordine del giorno così com'era stato formulato inizialmente.

con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di attribuire, al sistema nazionale, compatibilmente con la normativa europea e internazionale, anche funzioni di supporto tecnico allo allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione sull'impatto ambientale che i singoli prodotti nonché i materiali che li compongono hanno sull'ambiente». «impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché sia reso pubblico periodicamente sul sito ufficiale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale l'aggiornamento dei dati e delle informazioni statistiche di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica». PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, accoglie la riformulazione? Presidente, ho delle perplessità perché, così come viene riformulato, questo ordine del giorno non fa che ribadire quelli che già sono gli obblighi di legge sulla trasparenza e sulla diffusione dei

ulteriore noi lo accettiamo anche, ma questo è veramente far finta di voler prendere impegni, dobbiamo essere coscienti di questo. Non mi sembra che ci sia veramente la volontà del Governo di fare la differenza.

temporale perché quei fondi possano essere stanziato. Chiedo al Governo un ulteriore sforzo per provare a dare un impegno certo.

su richiesta della senatrice Moronese è stata valutata una proposta di riformulazione e, tuttavia, proprio per la particolarità dell'oggetto di questo ordine del giorno rispetto ad un provvedimento di carattere generale, il parere rimane contrario.

specificando cos'è il Sistema nazionale, dicendo che è istituito «al fine di assicurare l'omogeneità ed efficacia dell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di

«redazione di convenzioni con enti pubblici competenti in campo ambientale per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo

da parte di chi è stato demandato, in questo caso dallo Stato, a svolgere questo tipo di attività. Quindi sarebbe opportuno supportare questo emendamento che nulla toglie, non è politico, ma è semplicemente di buonsenso per dare efficacia all'azione legislativa.

non voglio approfittare del parere favorevole sull'ordine del giorno G3.103, sul quale ho insistito perché venisse rimossa la riformulazione, tuttavia l'emendamento 3.17 tratta lo stesso aspetto, ovvero prevede che il Sistema nazionale a rete debba anche effettuare, oltre all'attività di monitoraggio, che - lo ripeto - sulle opere infrastrutturali compete direttamente ai privati, anche la verifica della sua corretta esecuzione.

non può essere valutato sull'istante, in maniera statica, ma è un processo che dura una vita, quindi bisogna fare una valutazione anche dell'attività lungo tutto al Sistema nazionale delle Agenzie ambientali, credo che sia nelle definizioni, sia nelle applicazioni

Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per esprimere tutto il mio rammarico per quanto successo su questo giorno, sia per le modalità che per il parere contrario. le modalità, un attimo prima del parere del relatore, mi era stata consegnata una riformulazione. Vorrei ringraziare il sottosegretario Degani, perché c'è stato uno scambio

ero convinta del parere contrario sul primo punto e lo avevo detto anche nell'illustrazione, perché era impossibile avere il parere favorevole da parte di un Governo che, a quanto pare, è a favore di tutte le *lobby* che inquinano il nostro Paese,

per Costituzione, deve garantire la tutela della salute e dell'ambiente e non valutare se c'è questa possibilità.

per altri conflitti di interesse, forse si potrebbero impiegare gli stessi soldi per tutelare l'ambiente e la salute. Fatevi un esame di coscienza, perché questa contrarietà a quest'ordine del giorno è una vergogna! E io mi vergogno per voi!

propongono di dare all'ISPRA uno *status* giuridico di ente pubblico nazionale di ricerca, *status* che riteniamo assolutamente fondamentale, proprio all'interno delle funzioni di coordinamento del nuovo Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. È vero che nel testo si parla di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia

Il comma 4, che io propongo di sopprimere, attribuisce all'ISPRA il compito di adottare, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale a rete per

L'altro emendamento che vorrei brevemente illustrare e il 4.13,

è persona giuridica di diritto pubblico soggetta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e che l'articolo 7 stabilisce che le Agenzie regionali

impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire, anche tramite ulteriori strumenti normativi, al fine di garantire che le attività di ISPRA siano svolte in modo compatibile

8.3. L'articolo 8 si occupa di come vengono nominati i dirigenti generali e i direttori dell'ISPRA. Con questo Sistema nazionale a rete delle Agenzie ambientali

l'indipendenza dalla politica debba essere sancita anche e soprattutto dalle modalità con le quali vengono scelti i soggetti facenti parte di questo istituto. Chiediamo che sia per quanto riguarda l'ISPRA che per quanto riguarda le Agenzie, i soggetti vengano scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami tra professori, ricercatori universitari e il personale dell'amministrazione pubblica, per titoli, per competenze. Abbiamo anche presentato un ordine del giorno in tal senso, ma riteniamo estremamente importante

dall'articolo il termine «organizzativi» perché con riferimento ai LEPTA riteniamo imprescindibile che l'organizzazione debba continuare a dipendere dalle decisioni delle singole Agenzie

modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di adattarli a particolari situazioni orografiche, climatiche, paesaggistiche o antropiche locali».

triennale delle attività delle ARPA, anche se è solo per garantire il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale, debba tener conto in maniera vincolante del parere delle Regioni, che controllano le attività delle ARPA stesse. Quindi riteniamo che non basti il parere chiesto dalle Regioni, ma che serva l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato.

Siamo favorevoli al sistema a rete dei laboratori accreditati, per un'uniformità e una certezza di dati su tutto il territorio nazionale, ma non vorremmo cadere nel pericolo che questi laboratori non rispondano tutti alla stessa metodologia e ai sistemi riconosciuti a livello europeo come metodi efficaci e ufficiali di riferimento. Ecco perché ci teniamo - avrei dovuto presentare anche un emendamento al riguardo, ma c'è un ordine del giorno - che questa necessità venga ribadita, perché è importante che non si dia adito ad un'arbitrarietà

Posto che il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale, riteniamo che il Governo, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della legge, debba assumere iniziative ai fini dell'adozione di un principio di rappresentatività territoriale ponderata dalle singole Regioni, ai fini della definizione del potere di voto delle Agenzie regionali e delle Province autonome. È vero che le Agenzie non sono organi elettivi, ma sono comunque rappresentativi delle Regioni.

intervengo per illustrare l'emendamento 13.3, che propone la soppressione della parola «vincolante», al comma 2 dell'articolo 13,

ambientale». Mi pare già esagerata e assolutamente fuorviante la definizione «vincolante» su provvedimenti del Governo, ma quel che non riesco a capire è - lo faccio presente alla relatrice, al Governo e alla maggioranza - quale sia la definizione di «atti aventi natura tecnica in materia ambientale». A mio modo di vedere, questo comma è assolutamente fuorviante, molto pericoloso ed evidenzia le criticità non risolte che questo provvedimento porta ancora con sé. Mi auguro che vi sia lo spazio per modificare qualcosa in questi termini.

l'articolo 14 riguarda il personale ispettivo delle Agenzie regionali che pone in capo all'ISPRA la definizione di un regolamento che si base solo sul principio del merito per individuare il personale ispettivo. A noi francamente questa previsione non piace affatto. Non è un merito, perché chi stabilisce

intervengo per illustrare l'emendamento 14.9. Soprattutto noi campani sappiamo quanto sia limitante il fatto che non ci siano nelle Agenzie ambientali ufficiali di polizia giudiziaria. Questo è un ruolo indispensabile soprattutto per coloro i quali svolgono funzioni e compiti ispettivi e di vigilanza. tutti i soggetti che nel proprio esercizio svolgono queste specifiche funzioni operino con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Ciò innanzitutto per dare una qualifica certa a questi

che sono i primi a subire e a poter valutare quali sono i veri impatti sui territori.

l'articolo 15 tocca le noti dolenti dell'*iter* di approvazione di questo disegno di legge.

le risorse necessarie per essere funzionale allo scopo.

in Commissione alla Camera è stata inserita, articolo per articolo, l'invarianza economica e finanziaria per tutte le funzioni.

un anno ha fatto ostruzionismo. E quando il Governo fa ostruzionismo riesce a tenere fermi i provvedimenti anche per più di un anno, a differenza di quanto queste povere ed inesperte opposizioni riescono a fare. Laddove, poi, il provvedimento è arrivato in Commissione, vi è entrato a gamba tesa con un nuovo articolo, il 17, che

dopo un'attesa di oltre anno, esso doveva essere approvato al Senato in via definitiva. avevamo valutato l'opportunità di presentare ordini del giorno e di licenziare il provvedimento così come era, ci vediamo costretti a rimarcare

a questo Sistema ambientale di protezione e monitoraggio neanche un euro. Questo è gravissimo. Noi abbiamo quindi presentato delle proposte opportune all'articolo 15. Ribadiamo la necessità di un Fondo nazionale ambiente e giustizia, che venga anche incrementato con importi pari a 100 milioni di euro annuì per

a coloro i quali continuano a imporre la loro legge contro l'ambiente e i territori. [DE

(così come già accolta in discussione dell'ordine del giorno G3.100): «impegna il Governo a dotare il Sistema nazionale di ulteriori risorse al fine di implementare nel miglior modo possibile su tutto il territorio nazionale

A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti del Liceo scientifico statale «Galeazzo Alessi» di Perugia, che stanno assistendo ai nostri lavori.

vi sono solo 67 elettori per la bellezza di 62 candidati. È un paradosso. Mi fa piacere un tale eccesso di democrazia,

quindi, siffatti paradossi. Quello che mi fa specie è che noi parlamentari dovremmo modificare la legge quando non funziona invece il Governo, che di tutto si occupa tranne che dei cittadini e delle problematiche, costringe i propri parlamentari al paradosso opposto, e cioè

preme rappresentare in Aula la seguente situazione: Electron Italia è un'azienda controllata al 100 per cento da Finmeccanica, ora denominata Leonardo, nella quale lavorano 68 che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi integrati di sicurezza fisica per infrastrutture di rilevante importanza, settore che fa parte del *core business* dell'attuale Finmeccanica *one company*. Tuttavia, da oltre dieci mesi, Finmeccanica ha iniziato un procedimento di cessione di Electron Italia che sta destando numerose preoccupazioni nei lavoratori.

una sola azienda, la quale non pare avere i requisiti per garantire un futuro ai lavoratori. Al di là delle valutazioni di opportunità imprenditoriale, che non spetta a noi giudicare, anche se l'operazione sembra comportare la perdita di un patrimonio di competenze nel campo della sicurezza fisica, che costituiscono una realtà unica in Finmeccanica, che preoccupa maggiormente sono le prospettive dei 68 dipendenti dell'attuale Electron Italia, con il rischio di competenze notevoli disperse, di di capitale umano che si depaupera a scapito dell'intero sistema industriale italiano. Quale sarà il destino di quei dipendenti? Considerato che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro deve continuare con il cessionario, per quale per quale motivo i lavoratori sono così preoccupati? Quali procedure sono state attivate per garantire che non si verifichino eventi ulteriori dopo la cessione che legittimerebbero il licenziamento? Quali accordi d'ingresso o di armonizzazione sono stati previsti per assicurare la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori? Signor Presidente, pongo all'Aula del Senato questi interrogativi affinché le maestranze abbiano certezza che le massime istituzioni del Paese li ascoltino.

legge sulla riforma dei parchi, sono stato presidente di parco e vice presidente della Federparchi. Credo sia importante che l'Assemblea del Senato e il mondo delle aree protette italiane si uniscano